momento storico. Pensate infatti che prima di oggi non si era mai dibattuto di vitalizi in un'Aula del Senato. È un fatto curioso: sui vitalizi si sono spesi fiumi di parole e di inchiostro, ma il Parlamento non ne aveva mai parlato pubblicamente; non si era mai discusso pubblicamente dei vitalizi, nonostante questo fosse uno dei temi più caldi fuori da questo palazzo. Siamo felici

e non deve essere del MoVimento 5 Stelle. È un risultato frutto del lavoro di tutti. Certo, sul tema della giustizia sociale,

insieme agli amici del PD e di LeU, per iniziare finalmente quel processo - speriamo - di recupero culturale, etico, deontologico, comportamentale così necessario al Paese. Qualcuno ha detto che siamo giustizialisti perché facciamo questo; noi invece cerchiamo semplicemente di richiamare le classi dirigenti al rispetto di quelle regole che anche i cittadini non è giustizialismo. Crediamo che i partiti non debbano aspettare la magistratura per allontanare le mele marce dalla politica. Crediamo che chi ha amministrato o amministra la cosa pubblica ed è indagato per corruzione

E non perché lo dice il MoVimento 5 Stelle, ma perché lo recita l'articolo 54 della Costituzione, che stabilisce che tutti i cittadini devono comportarsi secondo le regole del rispetto e dell'osservanza delle leggi. Disciplina e onore chi ha gestito la cosa pubblica non sono a scadenza temporale; ci devono essere disciplina e onore in un parlamentare anche quando questi diventa un ex parlamentare, perché questa può essere la funzione del vitalizio. L'illegalità si può battere solo promuovendo il grado di maturazione civile dei cittadini. L'esempio, però, senatrici e senatori, deve partire da qui,

a tutela del prestigio e della credibilità delle istituzioni. Con la mozione presentata insieme agli amici del PD e di LeU chiederemo ai senatori e alle senatrici più pensioni e meno vitalizi. Chiederemo che si applichino ai vitalizi i principi della legge Severino, passaggio obbligato

e un vitalizio, perché non c'è un lavoratore italiano che possa percepire una pensione, dopo aver maturato quattro anni, sei mesi e un giorno: questo non è corretto.

indicazione nella nostra attività il contenuto della Costituzione, che non possiamo buttare alle ortiche. È prevista la cosiddetta autodichia

che non si è più d'accordo, allora aboliamo l'autodichia e mandiamo tutto ai tribunali ordinari. Finché l'autodichia esiste, non possiamo però buttarla alle ortiche.

La mozione che abbiamo presentato si pone solo un obiettivo, che non è quello di discutere o di annullare decisioni giurisdizionali passate in giudicato, perché non lo possiamo fare. Credo che sia evidentemente arrivato il momento di prendere in mano questa materia e, come è scritto nel dispositivo della nostra mozione, di affrontare una volta per tutte il problema nelle sedi competenti disciplinando quei casi - saranno individuati e indicati in maniera chiara - in cui si renda necessaria la revisione o la revoca del vitalizio verso quei senatori che siano cessati dal mandato e che siano stati condannati in via definitiva per reati particolarmente gravi.

Commissione contenziosa e Consiglio di garanzia sono organi giurisdizionali con tutti i poteri di un tribunale e di una corte d'appello, pertanto non siamo sicuramente in condizioni di metterli in discussione o di annullarli.

Signor Presidente, quando ho avuto notizia che un Gruppo parlamentare stava chiedendo di calendarizzare una discussione sui vitalizi sono rimasto basito, perché c'è ancora una camera di consiglio in atto che deve decidere sul famoso appello dell'amministrazione avverso la sentenza di primo grado che ha annullato la famosa delibera del 2018. Poi però ho letto le mozioni, che parlano sostanzialmente del vitalizio ai condannati, e mi ha fatto piacere che si sia aperta questa discussione, quantomeno per portare fuori da queste Aule ai cittadini un'informazione corretta su quanto sta succedendo. Mi auguro che i mezzi di informazione che seguono tale questione possano veicolare correttamente il dibattito che quest'oggi si svilupperà in Aula.

non deve soltanto applicare la legge ordinaria e la legge interna, ma la deve conformare ai principi costituzionali, perché l'autodichia ha escluso la possibilità per il parlamentare o per l'ex parlamentare di rivolgersi alla Corte costituzionale. pertanto gli organi di autodichia che, nell'espletamento della loro funzione, devono verificare se la norma che si impugna sia conforme anche alla Costituzione. Che cosa è successo? Ne possiamo parlare, perché le motivazioni sono state depositate. I titoloni dei giornali che vi tengono il velo: durante la notte sono stati ridati i vitalizi ai condannati; il Consiglio di garanzia ha ribaltato la decisione del Consiglio di Presidenza. quella decisione del Consiglio di Presidenza era incostituzionale, perché viola, presidente Licheri, non soltanto l'articolo 54, ma anche l'articolo 3 della Costituzione, secondo il quale tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. Dovete sapere - se non lo sapete che nell'esercizio della nostra funzione noi abbiamo fotografato il quadro normativo, costituzionale e ordinario, e siamo partiti dall'articolo 28 del codice penale, che stabilisce la sospensione di qualunque forma di assistenza, di vitalizio e di stipendio per i condannati che hanno avuto l'interdizione dai pubblici uffici: è il caso del senatore Formigoni.

e la n. 78 del 1967, secondo le quali non è sufficiente la semplice condanna o la semplice interdizione dai pubblici uffici per perdere un vitalizio, una pensione, un assegno, uno stipendio, ma si deve guardare alla gravità del fatto,

l'articolo 18*-bis* del decreto-legge n. 4 del 2019 - ancorché i vostri commentatori in televisione dicano di aver parlato soltanto del reddito di cittadinanza - prevede che ai soggetti condannati a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per reati gravissimi sia sospesa la pensione. Questa legge, presidente Licheri, io non l'ho votata. Io ho votato contro, l'avete votata voi. *(Applausi)*. Tuttavia, nel rispetto della mia funzione giurisdizionale, io ne ho dovuto tenere conto. Allora, Presidente, chiudiamo la partita. Se leggete la sentenza, noi abbiamo detto esattamente quello che avete chiesto voi: abbiamo detto che a un parlamentare o a un ex parlamentare deve essere chiesto un grado di onorabilità rafforzato rispetto al cittadino e se questo parlamentare o ex parlamentare ha sbagliato deve essere sanzionato; la sanzione deve essere stabilita dal Consiglio di Presidenza, ma nello stabilire la sanzione si deve tenere conto della gravità del reato e del rispetto della vita e della dignità umana (perché noi siamo un organo civile, non siamo dei barbari).

E consentite ai parlamentari e agli ex parlamentari di andare di fronte alla Corte costituzionale, così togliamo il disturbo presso gli organi di autodichia e ci rimettiamo dinanzi alla giustizia ordinaria. Anche questo è un esempio di parità tra cittadini e parlamentari.

approda in Assemblea - e per la prima volta - un dibattito sui vitalizi; un dibattito al quale, però, come riscontro osservando l'Aula, si sono sottratte molte forze politiche. Questo denota fondamentalmente un fatto molto concreto, che si vive anche fuori.

che si era condotta fino a quel momento secondo certi parametri. Insomma, è stato rivoluzionato tutto quanto. L'Italia stringe i denti, le persone ci guardano e l'esempio che dà il Senato in questo frangente è di assenza o di travisamento della realtà. *(Applausi)*.

il Parlamento, dandosi delle proprie regole in nome dell'autodichia e distorcendo questo principio, che rivendica la separazione dei poteri, si è auto attribuito privilegi, stipendi e vitalizi fuori dal normale, fuori dal contesto che vivono le persone. che vivono le persone. Nel 2018 arriva il MoVimento 5 Stelle e dice che, invece, come per le altre persone, vale il principio del sistema contributivo e non retributivo. È la grande rivoluzione che abbiamo portato in quest'Aula e che a giorni (anche questa) verrà sovvertita in nome della restaurazione. Si parla di diritto, ma vi sembra giusto che, dopo qualche giorno di legislatura, un senatore o un deputato, con un'integrazione, possa usufruire del vitalizio? Vi sembra normale che chi si attribuisce questi vitalizi poi lo faccia con le modalità più assurde, proprio in nome di questo privilegio? E poi, non contento di quanto stabilisce la legge Severino, che in altri casi prevede l'incandidabilità e l'ineleggibilità, prevede adesso che anche a chi sia stato condannato per corruzione o per gravi reati debba essere corrisposto il vitalizio. È una follia! *(Applausi)*. State parlando di qualcosa che è su Marte. Le persone guardano a questo dibattito con preoccupazione.

con il Paese. Con che coraggio continuate a dire di dare sostegni quando vi autoattribuite stipendi di migliaia e migliaia di euro e vitalizi? Fate come il MoVimento 5 Stelle: riducetevi le indennità e rinunciate a tutto ciò che è privilegio, che sovrasta il discorso che fuori di qui è molto sentito. È un dibattito che si può anche essere predisposti a sentire per le ragioni che vengono addotte, ma che è surreale. Ogni tassello, ogni parola che aggiungete a questo scempio e vergogna diventa un insulto ancora più forte fuori

della disattenzione o stanchezza delle persone che sono prese da altri problemi. E questo è ancora più grave. Vorrei sapere perché,

i Regolamenti, perché oltretutto considero anche opportuno che venga fatta una valutazione di caso in caso. Ho infatti difficoltà oggettivamente a pensare che possiamo privare del sostentamento una persona che vive in condizioni di indigenza totale in un sistema nel quale un condannato per reati gravissimi, come può essere l'omicidio o qualsiasi altro reato, continua serenamente a godere della propria pensione, dei propri emolumenti per sopravvivere. Ciò maggiormente in un sistema che ha introdotto degli istituti che sono quantomeno strani, se è vero come è vero (la cronaca è piena di esempi), che talvolta dei condannati per fatti gravissimi hanno goduto del reddito di cittadinanza. Allora qualche problema, qualcosa che non funziona evidentemente nel sistema c'è *(Applausi)* e dobbiamo prenderlo in mano. Discutiamone, proviamo a vedere come bisogna regolamentare questa materia una volta per tutte. Proviamoci, perché effettivamente ormai il tema è stato sollevato, con una ondata di populismo che francamente non condivido, perché a mio parere siamo qui per fare cose concrete,

non contestiamo quello che è previsto dalla Costituzione; eventualmente cambiamo le norme e i regolamenti. Eventualmente, se si pensa in un certo modo e la maggioranza richiesta dal Parlamento lo ritiene, potrà anche cambiare la Costituzione, ma fino a quando le norme sono quelle attuali, noi abbiamo il dovere, anzi l'obbligo, di rispettarle perché, come ho detto in molte circostanze, per me viene prima la Costituzione, poi tutto il resto.

il tema dei vitalizi è certamente molto delicato e trovo singolare che si debba discutere in quest'Aula di una decisione del Consiglio di garanzia che, come altri colleghi hanno già ricordato, è un organo giurisdizionale. Tuttavia, poiché il senatore Vitali e altri sono entrati nel merito, permettete anche a me di farlo, anche se sono un componente del Consiglio di garanzia, quindi forse mi perdonerete l'ineleganza di entrare nel merito di una decisione che ho contribuito a formare, anche se non sono stato d'accordo sulle conclusioni raggiunte con quella sentenza. Infatti, il presidente Vitali ha fatto dei riferimenti che, secondo il mio modestissimo avviso non solo di politico ma anche di modesto studioso di diritto, non mi convincono,

non risolvono la questione, perché entrambe fanno riferimento a pensioni derivanti da rapporto di lavoro,

Allora, cari colleghi, c'è qualcuno in quest'Aula che in buona fede può ritenere che noi abbiamo un rapporto di lavoro con il Senato della Repubblica? Siamo a busta paga? Abbiamo un salario? Abbiamo uno stipendio? O non abbiamo piuttosto un'indennità, che è tutta un'altra cosa?

era e rimane legittima. Rispetto il voto dei colleghi che, nel Consiglio di garanzia, l'hanno ritenuta illegittima, ma, a mio parere, il richiamo all'articolo 18-*bis* della legge n. 4 del 2019, cui faceva riferimento anche prima il senatore Vitali, non è pertinente:

per chi si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena e limitatamente a quel periodo; non ha nulla a che vedere con la questione di cui ci stiamo occupando e tantomeno

l'indennità di disoccupazione, l'assegno sociale, la pensione sociale e la pensione di invalidità. Non mi pare che si parli nemmeno di pensione. Badate bene, cari colleghi, non ha rilievo in questa sede nemmeno la dibattuta questione se il vitalizio abbia, in tutto o in parte, anche - come afferma la Corte costituzionale - una funzione previdenziale. Non è questo il tema, perché anche un'assicurazione privata può avere una funzione previdenziale. Il tema è se il vitalizio si fonda su un rapporto di lavoro o no,

Vitali. Questa è la ragione per cui voteremo a favore di tutte e tre le mozioni che sono state presentate oggi.

all'impegno di onore che ha assunto nei confronti del popolo italiano e delle istituzioni di svolgere con onore e disciplina la sua funzione abbia ancora diritto a ricevere un compenso, dopo aver tradito quell'impegno. Il vitalizio è una forma di indennità differita, proprio per garantire l'indipendenza e la libertà del parlamentare, che non deve avere preoccupazioni economiche. Un parlamentare prende un'indennità ragionevole, più che ragionevole. Ha fondi spesi a propria disposizione, uffici, servizi; ha una tranquillità economica, perché comunque sa che al termine del suo mandato potrà ottenere il vitalizio. Non ha alcun motivo e alcuna ragione di violare la legge per interesse personale privato, di suoi amici o di suoi conoscenti e nemmeno del partito. *(Applausi)*. Non c'è alcuna giustificazione per chi tradisce un impegno di onore come quello che tutti noi abbiamo assunto, in ragione della Costituzione sulla quale tutti noi abbiamo giurato. E allora qui non parliamo dei vitalizi in generale, ma parliamo dei vitalizi di chi ha tradito questo impegno. impegno. Siamo convinti che si debba andare nella direzione di fare una nuova delibera che rispetti questi principi; in questo senso, siamo qui e ci stiamo fino in fondo. Mi consenta, signor Presidente, solo un'ultima considerazione. Certo, collega Cucca, l'autodichia è una prerogativa costituzionale degli organi costituzionali; ritengo profondamente sbagliato però che ne facciano parte senatori, quando devono giudicare su questioni che riguardano i senatori. Nella Commissione contenziosa almeno abbiamo due esperti, mentre nel Consiglio di garanzia siamo cinque senatori. Caro Caro Presidente, credo che, quando si giudica di questioni e di diritti che riguardano i senatori, bisognerebbe trovare una soluzione per cui a giudicare non siano senatori,

la delibera n. 57, certamente non contribuisce a creare quella credibilità nell'opinione pubblica di cui oggi le istituzioni hanno tanto bisogno. *(Applausi)*.

alla lunga discussione che abbiamo avuto modo di fare in tema di prerogative parlamentari, sia ieri sia nei giorni precedenti. Giustamente, stiamo discutendo dell'onorabilità, dell'autorevolezza e della dignità del Parlamento. Vorrei fare una premessa: oggi in tutte le tre mozioni - ma parlo naturalmente per quella sottoscritta e promossa dal mio Gruppo - partiamo dalla premessa che c'è un regime di autodichia e che quindi prendiamo atto che c'è un vuoto normativo, conseguente a una pronuncia che non ha deciso solo sul caso specifico, ma che ha efficacia *erga omnes*. Ne prendiamo atto, sappiamo che c'è un vuoto normativo e crediamo che il Parlamento, nelle sedi opportune (che possono essere sia il Consiglio di Presidenza, sia una sede legislativa, perché su questo il Consiglio di Stato è stato chiarissimo, anche se ovviamente le conseguenze sono poi diverse, com'è stato già detto), il dovere di riproporre una decisione che tenga eventualmente conto, alla lettura, delle motivazioni che abbiamo già visto e che rileggeremo. La prima questione che rispettiamo assolutamente l'autodichia del Parlamento, ma anche il nostro ruolo, al quale non possiamo ovviamente venire meno.

Se non pensiamo e non sappiamo che è esattamente solo per questo che abbiamo prerogative e non privilegi, non diamo un indirizzo giusto e soprattutto, visto che parliamo sempre di ciò e di ciò che sta fuori di qui, non abbiamo titolo di parlare a chi sta fuori di qui e di cui incidentalmente siamo i rappresentanti, e non è che siamo stati designati.

diamoci pace: è pacifico che è una natura mista, che non può essere assimilata a un rapporto di lavoro e che ha natura anche previdenziale. I costituzionalisti si sono molto esercitati e gli atti sono tutti consultabili.

quella di chi è dipendente di un'amministrazione pubblica, quindi ha particolari doveri ed è anche destinatario di particolari norme incriminatrici. Sappiamo tutti che chi esercita un pubblico esercizio, è un dipendente pubblico e ha una pubblica funzione è destinatario di norme particolari. È qualcosa di molto di più: ma allora questo qualcosa di molto di più lo vogliamo inquadrare in un discorso complessivo che vale sempre e comunque? Vogliamo dire che siamo qui in una democrazia rappresentativa a rappresentare un'altissima funzione? È soltanto per questo motivo che abbiamo delle prerogative, a difesa della libertà del Parlamento, perché non è un caso che la Costituzione sia nata all'uscita dal fascismo, quando c'erano i tribunali speciali e chi dissentiva veniva messo in carcere. La prerogativa è nata esattamente con quel tipo di funzione e in quel senso,

Se è qualcosa di più e se dobbiamo stare dentro la Costituzione, che spesso viene richiamata nell'architettura costituzionale e non è semplicemente un'elegante

ci mettono in una situazione continua di ricerca di equilibrio tra beni costituzionalmente protetti. C'è l'articolo 54,

una direzione, da questo punto di vista, nel dover poi riformulare o ripensare una normativa, nelle sedi che riterremo (potrebbe essere il Consiglio di Presidenza, che è una sede legislativa). Sicuramente si può

parlando, ed è in questo che ci richiamiamo alla Costituzione, alle sue libertà e al suo inquadramento. Da questo punto di vista, la normativa andrà riscritta, tenendo anche conto di quei casi particolari in cui ci sono questioni umanitarie, particolari condizioni di salute o quant'altro,

cominciamo infatti anche a spogliarci di alcune immagini. Non è che qui c'è un palazzo chiuso e fuori un popolo pulsante, perché, mentre diciamo questo, stiamo svilendo la nostra funzione.

nel dire che è nel nome di tutti questi principi che pensiamo che ci sia una delibera ispirata alla questione dell'incandidabilità e di quant'altro; è nel nome delle cose importanti che facciamo al servizio dei cittadini che pensiamo che si debba fare quello; è nel nome di una coerenza con tutti i principi stabiliti nella Costituzione

non delle mani libere per tutti, ma di prerogative a difesa della democrazia. Noi siamo qui al servizio della democrazia liberale, quel trattino che non andrebbe mai dimenticato.

la delibera del Consiglio di Presidenza del Senato n. 57 del 2015, che prevedeva la cessazione dell'erogazione del vitalizio per gli ex Senatori condannati in via definitiva per reati gravi, e poi successive e contrastanti decisioni degli organi di autodichia del Senato, sino alla recente pronuncia del Consiglio di garanzia, che ha sostanzialmente annullato la suddetta delibera sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza, di cui all'articolo 3 della Costituzione, in relazione alla normativa sul reddito di cittadinanza. Il mandato parlamentare, essendo di natura elettiva, non è affatto assimilabile a un rapporto di lavoro. L'indennità parlamentare non può essere dunque qualificata come retribuzione, tanto che viene percepita per il solo fatto di ricoprire la carica, anche nel caso in cui il parlamentare si astenga da qualsiasi attività parlamentare, e serve ad assicurare l'indipendenza della funzione. Pertanto, il vitalizio, come proiezione dell'indennità, non può assolutamente avere natura previdenziale di retribuzione differita. La giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, così come la dottrina, hanno evidenziato la natura complessa e articolata dell'assegno vitalizio spettante ai parlamentari cessati dal mandato, che rappresenta un *unicum* specifico e particolare non riconducibile al trattamento previdenziale, non potendo avere alcun rilievo nemmeno il discrezionale mutamento del mero *nomen iuris* da parte delle Camere, che hanno recentemente cambiato in «pensione» l'originaria denominazione di «vitalizio», senza però che ciò ne abbia fatto mutare la natura giuridica. Peraltro, non sussistendo alcuna riserva di legge in materia di vitalizi analoga a quella prevista per l'indennità dall'articolo 69 della Costituzione, secondo il quale ad ogni membro del Parlamento spetta un'indennità stabilita dalla legge, poiché la Costituzione non menziona i vitalizi, non vi è dunque un diritto intangibile del parlamentare al vitalizio. Si tratta di un diritto costituito dal Consiglio di Presidenza, che ben può legittimamente escluderlo o limitarlo in casi specifici per il cadere di requisiti e condizioni che lo stesso Consiglio di Presidenza può porre. Allo stesso modo, gli organi di autodichia non potevano porre a raffronto, ai fini dell'affermazione del principio di uguaglianza, la norma sui vitalizi dei senatori con la disciplina prevista nei casi di condanna per gravi reati dalle norme sul reddito di cittadinanza, che sono funzionali a integrare il reddito familiare in attesa di trovare un lavoro e a contrastare la povertà e le diseguaglianze. La materia dei vitalizi è stata sempre disciplinata dai Regolamenti parlamentari, che hanno del tutto discrezionalmente creato il vitalizio e nessuno può mettere quindi in discussione che rimane una prerogativa dei Consigli di Presidenza delle Camere quella di modificare questa materia che essi stessi, con opera creativa, hanno costituito. D'altronde, vale un principio generale del diritto, oltre che di ragionevolezza, secondo il quale solo l'organo che produce una norma può modificarla. La Commissione contenziosa e il Consiglio di garanzia sono equiparabili, rispettivamente, ad organi giurisdizionali come il tribunale e la Corte di appello, in un sistema in cui i Regolamenti di Palazzo Madama hanno rango addirittura superiore, collocabile tra la legge ordinaria e la legge costituzionale. La delibera del Consiglio di Presidenza, quindi, ha lo stesso valore di una norma ordinamentale, come una legge, solo che, anziché limitarsi a decidere sul caso sottoposto al suo giudizio, l'organo giurisdizionale del Senato ha annullato la delibera *erga omnes*, cosa che può fare soltanto una contraria delibera di revoca da parte dello stesso organo che l'ha emessa. L'autodichia non può spingersi sino a consentire a un organo giurisdizionale come la Commissione contenziosa o il Consiglio di garanzia di annullare una delibera del Consiglio di Presidenza. È come se un giudice decidesse di abrogare una legge. Tuttalpiù avrebbe potuto decidere sul caso concreto con un'interpretazione della delibera costituzionalmente orientata o sospendere la decisione in attesa di una nuova pronuncia dell'Ufficio di Presidenza. Del resto, per motivare la decisione di primo grado si è fatto ricorso alla legge sul reddito di cittadinanza, con una sostanziale e riconosciuta equiparazione della delibera di un organo del Senato - badate bene - adottata da una sola Camera, a una legge bicamerale dello Stato, affermando che non è stato rispettato l'articolo 3 della Costituzione sull'uguaglianza dei cittadini. Mi chiedo allora: può un organismo interno al Senato dichiarare l'incostituzionalità di una norma **(ore 10,30)** (*Segue* GRASSO). Si possono addurre tutte le ragioni contrarie alla delibera del 2015, ma il riferimento che si è fatto in motivazione a due ordinanze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite non appare assolutamente coerente. Se si va a leggere, anche lì viene riconosciuto il carattere particolare dell'indennità parlamentare, da cui poi deriva, come proiezione, il vitalizio. Nel 2019 peraltro ci sono state decisioni della stessa Commissione presieduta dal collega Caliendo, citate nella sentenza, che sono state favorevoli a mantenere la delibera. Non sono riuscito a comprendere perché ci si sia discostati da quelle decisioni. Ripeto l'istanza oggetto della decisione l'ha presentata un singolo senatore e quella decisione avrebbe dovuto valere solo per lui. Consideriamo, però, anche le conseguenze: abolendo del tutto la delibera del 2015, si spalancano nuovamente le porte del vitalizio ai senatori condannati non solo per corruzione, ma anche per mafia e terrorismo. Spero proprio che non sia un effetto voluto, ma solo una distrazione. Per tutte queste motivazioni, giudico la decisione del Consiglio di Garanzia profondamente errata da un punto di vista procedurale, sostanziale e politico e ritengo che l'Assemblea, con la presente mozione, come organo politicamente sovrano, indurre l'Ufficio di Presidenza a intervenire adeguatamente per riaffermare le proprie prerogative decisionali in via definitiva. Sotto il profilo politico, inoltre, in un periodo in cui molti italiani sono in difficoltà, questa decisione investe uno dei temi che minano la fiducia del nostro sistema politico, che individuano le rappresentanze democratiche come casta e che allontanano ancor di più il Parlamento dai cittadini, e lo fa drammaticamente, proprio in un momento in cui, invece, dovremmo dimostrare l'esatto contrario. La condanna in via definitiva per determinati gravi reati è un mero presupposto oggettivo che determina una rilevanza così intensa sul piano del giudizio di indegnità morale del soggetto da esigere la cessazione dalle cariche elettive. questa conclusione vale se in gioco vi è non il diritto all'elettorato passivo, ma un assegno vitalizio. Il fondamento costituzionale è nell'articolo 48 della Costituzione. Il diritto di voto, attivo e passivo, a maggior ragione,

determinazioni, volte a disciplinare i casi di revoca dei vitalizi dei senatori cessati dal mandato condannati in via definitiva per delitti di particolare gravità, tenendo conto dei principi propri della normativa vigente in materia di incandidabilità, espressione della più generale categoria dell'ineleggibilità prevista dall'articolo 65 della Costituzione, valutando con rigore i comportamenti che appaiono incompatibili con quell'integrità morale che ci sforziamo quotidianamente di interpretare nella nostra funzione e che il Paese chiede a gran voce.

onorevoli colleghi, il tema dell'autonomia della politica e della sua funzione guida nella società, del suo non essere subalterna a poteri diversi e non sottoposti al controllo democratico, è un argomento del quale dovremmo molto interessarci, e non ricorrervi al bisogno, magari nelle interviste, nelle dichiarazioni televisive, nei *talk show* e nei comizi, per evocare poteri forti e oscuri che condizionano la vita pubblica e le scelte strategiche del Paese. Alcuni di voi potranno chiedersi cosa c'entri tutto ciò con i vitalizi. C'entra, eccome! La politica dell'ultimo ventennio e i parlamentari di quest'ultimo scorcio di vita repubblicana hanno genesi e storie politiche assai diverse da quelli del passato. Per tutto l'arco della prima Repubblica, la politica era una missione che caratterizzava in via esclusiva l'esistenza della vita di una persona, alla quale tutto era subordinato, ivi comprese le professioni e la stessa vita familiare. Con il tempo, questo percorso è cambiato; l'attività parlamentare è spesso accompagnata da altre e non rappresenta più un ostacolo per la professione. Questo, a mio avviso, è certamente frutto di un cambio di visione in cui la politica, ahimè, non è più centrale - circostanza che non gioca a favore della sua autonomia e del suo primato - ma è anche frutto dell'orda giacobina e del moralismo imperante che da oltre vent'anni si sono abbattuti sulla vita civile e democratica del Paese. Così il Parlamento e il parlamentare sono in balia di tutto, delegittimati dalle vulgate antipolitiche e sempre più privati non solo del ruolo di indirizzo, ma della stessa funzione legislativa. Questo è il risultato di una lunga stagione di demonizzazione della democrazia rappresentativa, nella quale abbiamo sostituito coloro che vivevano per la politica con l'improvvisazione e il dilettantismo e con alcuni che, sì, senza arte né parte, vivono oggi solo di politica e la usano per carriere e destini personali. Del resto, la perdita di competitività, prestigio e ruolo internazionale subita dall'Italia in questi anni è sotto gli occhi di tutti. È una deriva frutto della retorica contro la cosiddetta casta e dell'antipolitica che vede nel deputato e nel senatore un obiettivo da delegittimare, con argomenti che vanno dagli stipendi ai tanto odiati vitalizi. premessa: non cogliere la differente natura della pensione e del vitalizio dei parlamentari - spiegata anche in una sentenza della Corte costituzionale - dice già tutto di coloro che urlano e strepitano. È la Costituzione che ha voluto garantire all'esercizio della funzione parlamentare la massima libertà dai condizionamenti, anche di quelli di natura economica. Chi viola la Costituzione? Quelli che per anni hanno inneggiato all'intoccabilità della Costituzione più bella del mondo. Mi spiace poi contraddire ancora la retorica imperante: i parlamentari non possono in alcun modo essere equiparati ad alcunché, perché rivestono una funzione che non può essere paragonata ad alcun'altra funzione; svilirli non li renderà migliori e non ne aumenterà la produttività, la qualità e la rappresentatività. Certo, mi rendo conto che questa riflessione non sarà popolare, ma se non ribaltiamo il ragionamento andando oltre le convenienze del momento, distruggeremo definitivamente quel che resta del nostro sistema democratico e dei suoi istituti. Cos'era però l'istituto del vitalizio, se non una scelta per porre il politico in condizioni di indipendenza, libertà e autonomia? Attenzione, non solo l'indipendenza e l'autonomia dai poteri forti, ma dal lavoro e dal ricatto di non averne né trovarne uno, che costituisce una forma intrinseca di subalternità. Non c'è libertà, se si vive in una condizione di bisogno. Era una forma di garanzia di un'Italia che non c'è più, che forse è giusto in parte rivedere e superare. Infatti, gli interventi legislativi di questi anni, anche giustamente, hanno rivisto il tema dei vitalizi. Lo si è fatto con la mini riforma del 1997, poi nel 2007 e ancora nel 2012: siamo passati, seppur con le storture di applicazioni retroattive, da un metodo retributivo a uno contributivo. Ora qualcuno - magari proprio i professionisti della politica, quelli che vivono di politica e non per la politica, come diceva Weber o quelli che magari non hanno lavorato un solo giorno e votano qualsiasi provvedimento pur di non andare alle urne e lasciare, quindi, la tanto vilipesa poltrona vorrebbe pure abolirlo. Certo, si può ovviamente discutere su quale sia la misura congrua di indennità e di vitalizio atti a garantire al meglio la libertà di esercizio del mandato, ma considero offensivo, per la dignità di questa istituzione, che si usino parole come "ladri" che si appropriano indebitamente di risorse pubbliche, "scempio" o "vergogna". Sono parole indegne dei cittadini che rappresentiamo e della carica istituzionale che ricopriamo, che persino nell'uso del linguaggio ha il dovere dell'esempio. Dico no alla deriva e alle barbarie, come dico no all'accanimento e alla revoca del vitalizio a persone anziane o malate, che avevano fatto una previsione di vita per la loro vecchiaia su una base che non può essere stravolta, come difendo la delibera di questo ramo del Parlamento per far riavere il vitalizio, per ragioni di salute o di sussistenza, ad alcuni suoi *ex* membri. Occorre serietà: basta con la demagogia un tanto al chilo e con i moralisti che spesso si sono rivelati moralisti dei miei stivali. cari colleghi, l'ultimo anno ha cambiato il paradigma popolare, con l'emergenza che ha mostrato la necessità di una politica forte, capace di decidere, di governare e di progettare il futuro.

Lo facciamo non in nome di un qualche tecnicismo o espediente giuridico, ma della politica, della sacralità delle istituzioni repubblicane e della necessità di legittimazione dei suoi rappresentanti di ieri, di oggi e di domani,

il tema resta aperto e non ci sfugge, ma chi ha cultura di governo, sa vivere le istituzioni e crede nella democrazia e nei suoi presidi sa bene che ogni passo, per quanto piccolo sia, è sempre da considerarsi come una conquista.

che si ispirasse ai criteri messi in campo dalla Corte costituzionale, ossia la ragionevolezza e, dall'altra parte, il riferimento a un determinato periodo di tempo, chiaramente con la possibilità di reiterare eventualmente il provvedimento. Così la legge è stata votata dalla stragrande maggioranza di tutte le forze politiche

riferimento alla Corte costituzionale. Non capiamo - almeno non lo capisco io, poi magari qualcuno me lo spiegherà - per quale motivo si sia sempre voluto ricorrere all'altra possibilità per disciplinare questo argomento, ovvero ai cosiddetti regolamenti interni, interni, che inevitabilmente si prestano a ricorsi, su cui poi interviene il senatore, che deve giudicare su questioni legate ai senatori stessi.

quando iniziammo l'avventura con il Governo dei 5 Stelle. Gli dissi: «Guarda che la strada della legge è la migliore, perché ci consente di affrontare definitivamente il tema».

è una considerazione di carattere generale che sottopongo all'attenzione di tutta l'Assemblea, perché siamo sempre in tempo a fare una legge; non è che non possiamo farla. Passo alla questione della sentenza.

il riferimento alla sentenza della Corte costituzionale che equipara i vitalizi alle pensioni e il riferimento alla legge ordinaria sulla pensione e il reddito di cittadinanza. Non entro nel merito e non so se sia giusto o meno. Rispetto quella decisione; posso non condividerla, ma la rispetto per motivi appunto di rispetto nei confronti dell'istituzione e della sua autonomia. c'è qualcosa che stona in generale, indipendentemente dal fatto che si possa equiparare o no. A un cittadino condannato in via definitiva per terrorismo o per mafia non si può toccare o sospendere la pensione o il reddito di cittadinanza; ma se c'è un politico condannato, a lui bisogna per forza toglierla. *(Applausi)*.

con un'iniziativa tanti anni fa - io me la ricordo - denominata «zero privilegi», secondo cui i parlamentari non devono avere privilegi. È giusto e condivido il principio. Però, se è vero che i parlamentari non devono avere nessun privilegio anche in materia previdenziale, è anche giusto dall'altra parte che abbiano il diritto di non essere penalizzati sullo stesso argomento. *(Applausi)*. Si tratta semplicemente di mettere tutti sullo stesso piano. Del resto, quella delibera

e siamo assolutamente d'accordo nel lavorare in questa direzione, purché non si faccia sempre passare il politico come quello che sostanzialmente deve essere sbeffeggiato,

sbagliata - è la storia che ce lo insegna - è passare sempre da un estremo all'altro: prima i parlamentari erano troppo privilegiati, mentre adesso vogliamo farli passare come se fossero dei cittadini neanche di serie B ma, peggio ancora, come se fossero tutti dei ladri e dei delinquenti. la verità sta nel mezzo: recuperiamo il giusto mezzo, quello che storicamente ha nobilitato la politica in questo Paese. Solo così riusciremo a fare qualcosa di chiaro, che non possa più essere messo in discussione e che finalmente dia trasparenza e chiarezza su questo tema. Per questo motivo abbiamo presentato una mozione; non voteremo contro le altre mozioni, ci asterremo o voteremo a favore, a seconda della situazione, perché rispettiamo assolutamente tutte le posizioni (ci mancherebbe altro, anche perché la nostra mozione è quasi

per due settimane per poter avere semplicemente un confronto in Assemblea, che oggi, in base agli interventi svolti, mi sembra assolutamente costruttivo. Era un confronto necessario, visto che una norma che disciplinava che disciplinava la gestione dei vitalizi o, meglio, la revoca dei vitalizi per i condannati in via definitiva prima c'era; poi è intervenuta una sentenza che, andando oltre il *petitum*, l'ha e questo ha portato il MoVimento 5 Stelle a presentarsi in Conferenza dei Capigruppo per segnalare un vuoto normativo e la necessità di rimettere mano a ciò che stava accadendo. La prima reazione è stata voler fare una battaglia politica, di volerci appuntare la medaglietta, di voler portare di nuovo questo argomento, ormai abusato, all'attenzione dei cittadini. Devo dire che la mia prima reazione è stata quella di vergogna per chi pensava che la revoca dei vitalizi fosse esclusivamente una battaglia politica del MoVimento 5 Stelle: è una battaglia di dignità! *(Applausi)*. Dignità per il popolo italiano, senatore Romeo! È proprio per questa battaglia di dignità del popolo italiano che il MoVimento 5 Stelle nasce; nasce per la lotta contro i privilegi e contro la casta. A me sembra che, nello stesso momento in cui siamo stati esclusi da alcune caselle di questa che - è vero - non è una scatoletta di tonno, è un *bunker* antiatomico, che per poterlo scardinare non bastano otto anni, forse non ne basteranno venti; come siamo stati esclusi da qualche casella (la Commissione contenziosa e il Consiglio di garanzia), grazie al tradimento di nostri colleghi *(Applausi)*, eletti grazie alla fiducia ricevuta da parte di cittadini su un programma che si basava fondamentalmente sulla lotta alla casta e sul taglio ai vitalizi, miracolosamente, con un colpo di mano, abbiamo visto ripristinare i vitalizi ai condannati.

correttamente all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza. Avevamo visto la sua mozione, che era sinceramente irricevibile, però oggi ne presentate un'altra, dove si legge: «Impegna a rivalutare nelle sedi competenti, nel rispetto dei principi dell'articolo 54 della Costituzione».

di onorabilità e disciplina nell'aver usato la sanità pubblica della Regione Lombardia come fondo cassa per viaggi da sogno e *yacht* di lusso per sé e i suoi amichetti? *(Applausi)*. è stato condannato a risarcire 47 milioni di euro. Mi domando: adesso gli ridiamo il vitalizio così lui ci ridà i 47 milioni di euro?

Mi corre l'obbligo di ricordare alcuni nomi e reati, perché credo che oggi ci sia la possibilità di far capire anche ai cittadini italiani di chi e cosa parliamo. Parliamo dei senatori Berlusconi,

e, per poter riconoscere un privilegio a un corrotto, fate riferimento all'articolo 18-*bis* della legge sul reddito di cittadinanza. Le dico una cosa.

Oggi l'unico intento di questa mozione è far capire ai cittadini italiani cosa si pensa dei vitalizi ai condannati: se ritenete che una persona condannata per gravi reati abbia diritto a godere di un privilegio, oppure no.

il Consiglio di garanzia e l'Ufficio di Presidenza. Volevamo aprire questo luogo e apriamolo. Oggi dovete dire agli italiani se volete revocare i vitalizi ai condannati semplicissimo, rispetto a parole che devo leggere: la nostra posizione era e rimane coerente; sul taglio dei vitalizi faremo tutto quello che è possibile in un momento come questo, in cui ci sono famiglie a cui viene chiesto indietro l'assegno di accompagnamento per i figli disabili, in cui ci sono famiglie che non hanno visto la cassa integrazione, in cui ci sono famiglie che stanno perdendo il negozio e la speranza; il mancato taglio dei vitalizi è un segnale disgustoso e vergognoso. Queste sono le parole del senatore Salvini

Abbiamo iniziato questa battaglia alla Leopolda nel 2011, ora c'è da fare l'ultimo miglio e per me va fatto subito. Sono parole del

eravamo tutti d'accordo. Vanno tagliati i vitalizi ai condannati; i vitalizi vennero aboliti nel 2012 dal Centrodestra, fu una nostra iniziativa; lavoriamo da sempre per avere un sistema politico-istituzionale meno costoso e più efficiente, avevamo anche approvato una riforma costituzionale che riduceva il numero dei parlamentari, che però fu impedita dalla Sinistra. Tranquilli tutti, l'abbiamo fatta noi. Non mi sembra che questo sia il momento giusto per discutere di queste cose (invece questo sì, questo è il momento giusto). Siamo al lavoro per sostenere un Paese che soffre, non c'è tempo da perdere per parlare di vitalizi e di decisioni già prese. Questo lo ha detto il 27 giugno 2020 Silvio Berlusconi

Platone diceva che le brave persone non hanno bisogno di leggi che dicano loro di agire responsabilmente, mentre le cattive persone troveranno un modo per aggirare le leggi. Noi, brave persone, non torneremo indietro.

e anche di non fare fotografie, che è vietato a tutte le persone, brave o cattive che siano.

data la riconosciuta importanza della discussione da parte di tutti i Gruppi, cerchiamo di avere un comportamento conseguente. CALIENDO *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente,

non ha possibilità di parlare se non con atti. Pertanto io non interverrò sulla questione, perché abbiamo già fatto la sentenza, ma non voterò nessuna delle mozioni, in primo luogo perché nel 2011, quando chiesi di parlare su quel documento che era il regolamento sulle pensioni dei senatori, mi fu detto

il blocco per i pensionamenti anticipati. Lei sa benissimo che la sentenza Pagliari sulla certificazione, come avviene per i vitalizi, non può essere messa in discussione. No. Abbiamo affermato che i vitalizi sono una previdenza? No. Abbiamo preso atto che le sezioni unite della Corte di cassazione, ovvero l'organo che assicura l'uniforme applicazione del diritto del nostro Paese ha affermato che è un trattamento di natura previdenziale. Questo comporta l'applicazione delle regole della Corte costituzionale.

attraverso la piazza, le regole del processo e di imporre ai giudici di rispettare la volontà del popolo. Ringrazio la presidente Bernini e il presidente Berlusconi, perché su queste materie non ho dovuto mai discutere nel Gruppo e nel partito, né del calendario delle udienze, né di quali fossero i sistemi e le logiche. So che fate le riunioni di Gruppo sulle questioni giurisdizionali, siamo completamente fuori dalle regole di uno Stato democratico. *(Applausi)*. Il giudice decide secondo coscienza e secondo la legge.

Presidente, intervengo a maggior ragione dopo l'intervento del senatore Caliendo per evidenziare come le mozioni presentate contro il ripristino dei vitalizi per i parlamentari condannati non colgano la sostanza del problema e cioè che con la decisione presa è come se al Senato si fosse consumato una specie di *golpe*, anzi un auto *golpe*, con un conflitto di poteri tra organi interni che non ha precedenti nella storia della Repubblica. In materia di autodichia la Commissione contenziosa vale, come è noto, come un tribunale. Ebbene, la sentenza con la quale ha deciso di restituire il vitalizio al senatore Formigoni non si è limitata, come diceva il senatore Grasso, a giudicare su un caso specifico, ma ha addirittura proceduto ad annullare una delibera del Consiglio di Presidenza.

al suo intervento. Dico a tutti i colleghi senatori che più di uno non solo ha lambito, ma è arrivato anche a discutere nel merito della sentenza, ha iniziato prima il senatore Vitali e poi altri senatori intervenuti

ma, se si entra nel merito della decisione oltre un certo limite, questa Presidenza non lo consentirà,

Per questo credo ci siano i margini doverosi affinché il Senato sollevi di fronte alla Corte costituzionale un conflitto di attribuzione. L'invasione di campo di un organo giurisdizionale ha inflitto un *vulnus* al principio della separazione dei poteri e penso che il Consiglio di Presidenza abbia il dovere di promuovere questa iniziativa. Altrimenti - lo dico a tutti i componenti che ne contestano la decisione

dagli organi presieduti dai senatori Caliendo e Vitali. *(Applausi)*. Dirò di più, Presidente: c'è un'altra vergogna sulla quale questo Parlamento continua a tacere.

utilizzandone tutti i privilegi, mentre potrebbe cancellarla in cinque minuti con una delibera del Consiglio di Presidenza. È quella delle doppie e triple pensioni, accanto ai vitalizi, che i parlamentari continuano a lucrare a danno dei cittadini, grazie allo scandalo dei contributi figurativi.

Lo scandalo dei contributi figurativi. Come oggi ha ricordato l'ex presidente dell'INPS Boeri, ci sono centinaia di parlamentari

Rispetto a questo non possiamo rimanere inerti, perché, mentre in quest'Aula i senatori si concedono privilegi odiosi, fuori ci sono cittadini disperati, senza lavoro costretti a pagare la vergogna dei vitalizi e dei contributi figurativi.

Sì, Presidente, perché si parla di democrazia, ma si vuole imbavagliare il Parlamento. PRESIDENTE. Non si preoccupi che il Parlamento in questo momento è liberissimo.

la sentenza è stata pubblicata e, quindi, è pubblica. Sono stati fatti interventi sulla sentenza e, siccome sono il relatore della sentenza, intervengo in dissenso anche per questo motivo. Non farò un comizio, come altri, perché i comizi li faccio in campagna elettorale; né citerò casi personali politici, perché anche questi non appartengono al dibattito civile in quest'Aula. Voglio soltanto dire alla presidente Taverna che esiste l'articolo 57, ma esiste anche l'articolo 3 della Costituzione, per il quale ogni cittadino deve essere trattato alla stessa maniera

che consente ai condannati non per reati gravi di continuare a mantenere la pensione e l'assegno, non ho capito per quale motivo il parlamentare debba essere trattato in maniera peggiore di un qualunque cittadino. (*Commenti*). Fatemi parlare! Concludo parlare! Concludo perché mi aspetto che qualcuno chieda scusa per quegli *slogan*, chiaramente se c'è onestà intellettuale; se non c'è onestà intellettuale, ognuno fa ciò che vuole.

perché con la sentenza non è stato ridato il vitalizio ai condannati. Con la sentenza è stato stabilito che l'*ex* parlamentare deve avere un grado di onorabilità maggiore rispetto al cittadino e che le sanzioni vanno comminate dal legislatore interno (il Consiglio di Presidenza), ma tenuto conto dei principi di ragionevolezza stabiliti dalla Costituzione, come per tutti i cittadini, per garantire il rispetto della dignità e dei diritti umani. Questo dice la sentenza e questo è praticamente ciò che chiedono le mozioni. Per questo motivo voterò in dissenso.

i vitalizi a coloro che sono stati condannati. Leggetele; sono pressoché identiche e, tuttavia, i vitalizi sono stati restituiti a coloro che sono stati condannati per gravissimi reati. Allora, ai partiti presenti e, soprattutto, a chi sventola cartelli con la scritta «no ai vitalizi» dico che avete un modo specifico per far per far cessare tutto ciò: staccate la spina al Governo e fate andare a casa questa maggioranza indecente. Altrimenti, la sensazione è che queste mozioni e questi piagnistei siano un mero lavaggio delle coscienze. A questo L'alternativa c'è non si presta e non voterà queste mozioni per i motivi che ha spiegato benissimo il collega Primo Di Nicola, in dissenso dal MoVimento 5 Stelle. *(Applausi)*.

Presidente, i cittadini capiscono una cosa: i condannati si riprendono il vitalizio. Questa è la cosa più facile che i cittadini hanno capito e che prenderanno. Quindi, è giusto che io dia il pieno sostegno alla mozione del MoVimento 5 Stelle, perché ho fatto la campagna elettorale su questi temi, moralmente importanti. Mi asterrò sulle altre due perché voglio riconoscere al Movimento un lavoro che è stato fatto da tempo. È proprio per questo che domando, in nome dell'etica e della morale, morale, attraverso la Presidenza al Movimento: perché ai condannati è giusto non dare il vitalizio, ma a un condannato per gravi reati finanziari, perché ha truccato i bilanci di Monte Paschi di Siena,

condannato in primo grado, è ancora amministratore delegato di una partecipata di Stato quotata in borsa? Perché il Movimento non gli toglie la fiducia? Perché non sollevate anche voi, attraverso il Governo, l'azione di responsabilità verso questo condannato per gravi reati finanziari? L'aspetto morale deve valere quindi per tutti. Sì dunque a questa mozione, sì all'aspetto etico che sollevate, ma basta con i condannati che guidano delle partecipate di Stato quotate in borsa.

Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 16, con la votazione per l'elezione di due senatori Segretari. *(La seduta, sospesa

Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento, ciascun senatore o senatrice scriverà sulla propria scheda un solo nominativo. Risulteranno eletti i due senatori che otterranno il maggior numero di voti. A parità di voti sarà eletto il più anziano di età. Per garantire il più ordinato svolgimento delle operazioni di voto, dinanzi al banco della Presidenza sono state approntate due cabine. I colleghi senatori, immediatamente prima dell'ingresso in cabina, riceveranno dagli assistenti parlamentari la scheda che, dopo il voto, depositeranno nell'apposita urna all'uscita della cabina stessa. La chiama sarà svolta in ordine alfabetico. Dopo l'effettuazione della chiama, le urne resteranno aperte fino alle ore 19, mentre l'Assemblea proseguirà nell'esame del successivo punto all'ordine del giorno. Dichiaro pertanto aperta la votazione e invito il senatore Segretario a procedere all'appello.

Di Girolamo,

Grazie a tutto

senatore Ferrara, Signor Presidente, l'intesa in esame è finalizzata a consolidare e approfondire ulteriormente la collaborazione tra i due Paesi nell'ambito della ricerca pubblica e privata in campo scientifico e tecnologico, già prevista per grandi linee dall'Accordo di cooperazione culturale bilaterale del 1975, nonché a migliorare le rispettive conoscenze tecnologiche e dotazioni infrastrutturali, anche a beneficio del mutuo sviluppo economico. Il disegno di legge di ratifica si compone di cinque articoli. L'articolo 3, in particolare, modificato dalla Camera dei deputati, quantifica gli oneri economici derivanti dalla cooperazione scientifica e tecnologica, di cui all'articolo IV dell'Accordo, in 461.000 euro annui a decorrere dal 2020 e le spese di missione dei funzionari dei reparti di cui all'articolo X in 7.200 euro ad anni alterni a decorrere dal 2020. L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese. In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Signor Presidente, nel dichiarare il voto favorevole per il Gruppo Italia Viva, chiedo l'autorizzazione a depositare il testo integrale dell'intervento.

si ricollega a un'intesa, già prevista, di delimitazione dei rispettivi spazi marittimi, che risale addirittura al 1977 e che è ancora vigente, con la quale i due Stati, Italia e Grecia, hanno delimitato la piattaforma continentale del Mar Ionio. Nessuno dei due Paesi - tengo a sottolineare al momento - ha proclamato aree di giurisdizione funzionale, sia come pesca riservata sia come zona di protezione ecologica o come zona esclusiva economica sulla colonna d'acqua del Mar Ionio. Tuttavia - mi preme ricordarlo - un apposito disegno di legge, l'Atto Senato 2007, già approvato dalla Camera dei deputati e attualmente all'esame della Commissione affari esteri del Senato, prevede espressamente l'istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale. Per quanto riguarda i profili di compatibilità con la normativa nazionale, anche quest'atto non presenta alcun tipo di problema. Propongo pertanto il voto favorevole dell'Assemblea.

Dichiaro chiusa la votazione

l'Assemblea è chiamata a votare questo provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, per permettere all'Ecuador di aderire a un Accordo già in essere fra

Il testo in esame costituisce lo strumento giuridico con cui l'Ecuador aderisce all'Accordo multipartito sottoscritto nel 2012 dall'Unione europea e dai suoi Stati membri con Colombia e Perù, e cioè al primo Accordo commerciale concluso dall'Unione europea dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che rappresenta un importante strumento per la crescita e lo sviluppo dell'integrazione regionale fra Europa e America Latina, che permette di rafforzare i legami politici ed economici tra le due aree geografiche. Tra gli aspetti di rilievo posti in evidenza nella relazione, che accompagna il disegno di legge di ratifica, la valutazione della Commissione europea circa gli aspetti attesi con l'adesione al protocollo, che dovrebbe consentire un aumento delle esportazioni dell'Unione europea verso l'Ecuador per cento; un risparmio di dazi per gli esportatori dell'Unione europea nella misura di almeno 106 milioni di euro l'anno e nuove possibilità di accesso al mercato per quanto riguarda i prodotti del settore agricolo, dell'*automotive* e dei macchinari. Il disegno di legge di ratifica del Protocollo si compone di quattro articoli e l'articolo 3 pone in particolare una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'analisi della compatibilità dell'intervento non segnala criticità dal punto di vista dell'ordine costituzionale, né di contrasto con il diritto europeo e con altre norme di diritto internazionale a cui l'Italia è vincolata.

del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e Atto finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996,

Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica degli emendamenti all'Accordo del 1996 sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua. L'Accordo costituisce uno dei principali strumenti giuridici internazionali finalizzati alla conservazione della biodiversità e a ridurre le minacce a carico della sopravvivenza dei cetacei in quelle acque. Il provvedimento prevede anche la creazione di una rete di aree marine protette e la regolamentazione delle attività di pesca dei cetacei. Il disegno di legge di ratifica pone una clausola di invarianza finanziaria; stabilisce che dall'attuazione della ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate debbano svolgere le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali ed è per questo che, in qualità di relatrice, propongo l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea. *(Applausi)*.

ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013

La relatrice, senatrice Rojc, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi recante la ratifica dell'Accordo tra Italia e Kirghizistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, sottoscritto nel febbraio 2013, rinnovando l'ultima Intesa relativa a tali ambiti risalente addirittura al 1960, anno della firma dell'Accordo di cooperazione culturale tra Italia e Unione Sovietica. Scopo primario dell'Intesa è quello di migliorare la conoscenza e la comprensione tra i due popoli e promuovere i rispettivi patrimoni culturali attraverso lo scambio di esperienze e dati, soprattutto a livello scientifico e tecnologico, su basi paritarie e di reciprocità, fornendo nello stesso tempo una risposta efficace alla forte richiesta di cultura e lingua italiana in Kirghizistan. Si ricorda che l'Assemblea del Senato ebbe modo di esaminare e approvare il testo del presente disegno di legge, in prima lettura, il 30 ottobre 2019. Le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, conseguenti a un parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione formulato dalla Commissione bilancio, riguardano l'articolo 3 relativo alle disposizioni finanziarie della ratifica, e posticipano di due anni la relativa autorizzazione di spesa. Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di cinque articoli, con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento. L'articolo 3 li valuta in poco più di 135.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, e in 139.620 euro a decorrere dal 2023. Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese e, quindi, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale. La relatrice, senatrice Craxi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi l'Assemblea è chiamata nuovamente a esaminare il disegno di legge, approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati, recante ratifica della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia, fatta a Riad, in Arabia Saudita, nel febbraio 2011. Si ricorda che l'Assemblea del Senato ebbe già modo di esaminare e approvare il testo del presente disegno di legge, in prima lettura, il 30 ottobre 2019. Le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, conseguenti a un parere favorevole con condizione, volto a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, formulato dalla Commissione bilancio, riguardano l'articolo 3, relativo alle disposizioni finanziarie della ratifica, e posticipano di due anni la relativa autorizzazione di spesa. Il disegno di legge di ratifica della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia si compone di quattro articoli. L'articolo 3, in particolare, valuta gli oneri economici complessivi del provvedimento, a decorrere dall'anno 2021, in 151.920 euro, di cui 51.920 euro annui per le spese di missione e 100.000 euro annui per il contributo finanziario obbligatorio. La ratifica della Carta non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese. In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea. *(Applausi)*.

Con impegno e grande senso di responsabilità, il Senato ha da poco istituito la Commissione di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati. L'iniziativa parlamentare testimonia la consapevolezza unanime che gli *standard* di sicurezza, benessere, garanzia, legalità ed equità degni di una democrazia avanzata come la nostra

e proiettati verso traguardi di civiltà, non possiamo ora permetterci un'inversione di marcia e ragionare, come sembra stia invece facendo il Governo, su provvedimenti che riporterebbero indietro il Paese di oltre mezzo secolo in termini di tutela. La prospettiva che il cosiddetto decreto semplificazioni ripristini il ricorso al criterio di aggiudicazione basato sul massimo ribasso ci allontana dall'obiettivo delle tutele e, soprattutto, dal traguardo auspicato di non dover più ricorrere in futuro a indagini pubbliche e pubbliche ammende sulle troppe storture che reprimono un diritto costituzionalmente riconosciuto. L'attuale codice degli appalti ha tradito nei fatti più di un'aspettativa di semplificazione e modernizzazione del Paese,

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il prossimo 12 giugno saranno trascorsi dieci anni dal *referendum* del 2011 che vide il popolo italiano esprimersi contro la privatizzazione del sistema idrico. Con il secondo quesito del *referendum,* nella determinazione della tariffa del servizio idrico integrato è stato abrogato, all'articolo 152 del codice ambientale, il riferimento all'adeguata remunerazione del capitale investito. Non sono bastati 26 milioni di sì, con oltre il 57 per cento degli aventi diritto che si è democraticamente espresso, per riuscire a trasformare il sistema idrico italiano, soprattutto in Regioni come la Campania, dove gestioni come quella della GORI continuano a vessare i cittadini con continui aumenti tariffari, disservizi e mancati investimenti. Quello dell'acqua pubblica è un tema importantissimo. Ci siamo sempre battuti per il principio dell'acqua come bene comune, indispensabile e accessibile a tutti senza distinzioni ed essenziale per la sopravvivenza. Per la ripubblicizzazione del sistema idrico esiste una proposta di legge ferma alla Camera dei deputati, presentata da quelli che erano i miei colleghi del MoVimento, nella quale sono ribaditi i principi generali dell'acqua come bene naturale, diritto universale, fondamentale e indispensabile per la vita. È intollerabile, dunque, che la volontà popolare non sia rispettata. In Campania il 98 per cento dei votanti si era espresso a favore del secondo quesito referendario. L'acqua è un bene pubblico e tale deve ritornare. Su questa posizione dobbiamo essere coerenti con la decisione referendaria. Non è possibile ancora oggi avere gestori come la GORI, che fanno dell'acqua un affare pagato dai cittadini a caro prezzo, con tariffe sempre più esorbitanti e allo stesso tempo non ci si pensa due volte a intimare o chiudere l'erogazione se non si è in grado di pagare bollette sempre più esose, frutto di rincari continui e ingiustificati. L'accesso all'acqua è un diritto umano universale ed è anche una condizione essenziale per arginare la drammatica emergenza igienico-sanitaria che stiamo vivendo. Ragionare su aumenti delle tariffe in un momento di crisi economica e sociale come quella che stiamo vivendo a causa dell'emergenza Covid, con famiglie ridotte sul lastrico e difficoltà crescenti per trovare un'occupazione, è veramente inammissibile. A dieci anni da quel *referendum,* ispirato da oltre 400.000 firme raccolte dai movimenti per l'acqua e confermato da milioni di italiani, non abbiamo ancora una rete di infrastrutture idriche degne di uno dei Paesi più sviluppati del mondo. Questo è gravissimo e sento oggi il dovere di sottolinearlo e di invitare tutti ad una riflessione su questo argomento

Si sono susseguiti più Governi, con maggioranze diverse, ma l'atteggiamento è rimasto sempre uguale: scarsissima attenzione alle voci che provengono dal territorio e che, attraverso i parlamentari, vogliono giungere fino all'Esecutivo. I cittadini aspettano risposte ed attenzione, invece devo riscontrare che ricevono soltanto indifferenza: ne sono la testimonianza. Tra le tante interrogazioni cui

periodo 2020/2021. L'Agenzia delle entrate sta applicando sanzioni ed interessi che, sommati, giungono a soglie di assoluto allarme, ben oltre il 100 per cento dell'imposta, a seguito della decadenza del beneficio del pagamento rateale. Tanti sono i contribuenti, persone fisiche e giuridiche, che non sono riusciti ad ottemperare ai pagamenti rateali verso il fisco a causa della pandemia, che ha determinato pesanti cali di liquidità per gli scarsi l'attivazione della cassa integrazione Covid. L'Agenzia delle entrate non può richiedere l'intero pagamento del debito, aggravato da interessi e sanzioni, nel termine giorni solo a seguito di un ritardato pagamento, a volte anche soltanto di una sola rata, e la conseguenziale decadenza dal beneficio del termine, data la straordinarietà della crisi economica in cui vive il Paese. Interessi e sanzioni così alti praticati dall'Agenzia delle entrate indeboliscono fortemente la battaglia che lo Stato conduce nella lotta all'usura, ritenendola un fenomeno da contrastare con forza. Per questo, proprio in questo momento di grave recessione economica, è necessario porre rimedio. Ho chiesto al Ministro di sapere le ragioni per cui il Governo non vigila attentamente sull'applicazione del tasso di interesse e sulle sanzioni applicate dall'Agenzia delle entrate che, secondo calcoli effettuati, supera il 100 di ricarico sull'imposta dovuta; se e quali iniziative di competenza il Ministro intenda inserire nei prossimi provvedimenti, al fine di determinare più eque condizioni di pagamento per coloro che sono decaduti dal beneficio della rateizzazione, della definizione agevolata o della rottamazione. Ho chiesto, inoltre, se non ritenga di assumere una decisione urgente per porre rimedio alla succitata condizione di squilibrio adottata dall'Agenzia delle entrate nei confronti dei contribuenti italiani. Queste Queste sono le domande che ho posto al Ministro e mi auguro che possano arrivare presto le risposte, non per me, ma per i cittadini. [BOSSI Signor Presidente, quelle che sto per leggere sono le parole di uno dei più importanti uomini che hanno reso e ancora oggi rendono la pesca sportiva italiana famosa nel mondo, più volte è stato premiato in ambito sportivo, è scrittore di libri e documentarista e quindi anche figura di riferimento per questo importante settore. Si chiama Roberto Ripamonti e mi scrive in merito a una problematica seria, quella delle reimmissioni: reimmissioni: «Caro Simone, come ben sai la pesca sportiva in Italia muove un dinamico ed importante tessuto sociale, culturale, sportivo e produttivo; è un importante vettore per portare i più giovani verso l'aria aperta, è svago per i più anziani, è sana e funzionale attività per i disabili. I praticanti sono più di due milioni, l'indotto supera i tre miliardi di euro e sono oltre 15.000 i lavoratori in tutto il settore. La pesca sportiva è anche uno strumento turistico e conseguentemente vettore economico di rilevante importanza per tutti i territori bagnati dai fiumi, dai laghi, dai torrenti spesso è l'unica vera attrattiva turistica a fronte di un indotto. In Nazioni limitrofe (Austria, Croazia, Bosnia e Slovenia) questa attività è strutturata e attira decine di migliaia di appassionati in tutta Europa per beneficiare delle acque gestite con criteri imprenditoriali ma rispettosi dell'ambiente naturale. I nostri corsi d'acqua sono oggetto di minacce che vanno dagli scarichi industriali al prelievo idrico al bracconaggio, per non parlare della mortale presenza di specie ittiofaghe quali il cormorano, vero distruttore di *stock* ittici dei torrenti. I ripopolamenti, quindi, sono l'unico vero strumento di ripristino degli equilibri. I ripopolamenti. L'adozione di criteri scientifici esattamente restrittivi ha bloccato l'immissione per scopi di ripopolamento nella quasi totalità del territorio nazionale, alterando un equilibrio gestionale raggiunto da oltre un secolo. Il decreto attuativo del 2 aprile 2020, con riferimento all'articolo 3 criteri per l'immissione in natura di specie o popolazioni non autoctone sta ottenendo risultati devastanti per l'intero settore per il blocco di immissioni della trota fario, della trota iridea e del coregone. Il perdurare delle minacce sopra descritte, a fronte di mancati ripopolamenti, ha svuotato i corsi d'acqua italiani, allontanando migliaia di appassionati con danni devastanti per le attività economiche collegate. È inoltre entrato in crisi un settore, quello della piscicoltura, che vede sottrarsi una importante fonte di fatturato senza la possibilità di predisporre adeguamenti al mutato quadro normativo. Migliaia di posti di lavoro sono quindi a rischio per una scelta superficiale, inopportuna ancor più in presenza di una pandemia. È necessario pertanto ripristinare le immissioni in ottemperanza delle esistenti carte ittiche, ignorate da questo decreto, ridisegnando un sistema normativo adeguato alla realtà mediante un documento che consenta con effetto immediato l'immissione di esemplari adulti e sterili delle specie alieutiche di interesse; tutto ciò al fine di ripristinare una situazione consolidata in oltre cento anni di immissioni e permettere a tutto l'indotto economico attualmente bloccato di ripartire. Con stima, Roberto». che qui si sta ammazzando un settore intero. Non è bastata la pandemia ad uccidere gli uomini e le attività. Da dove e per quale motivo arriva questa stupida volontà di distruggere un settore fatto di attività sane? Queste sono scelte ingiustificate. È troppo facile riempirsi la bocca al giorno d'oggi di belle parole come «ambientalismo», «ecologia», «salvaguardia dei corsi d'acqua». La realtà è che questa è solo stupida e miope ideologia estremista che non giova a nessuno, né all'ambiente, né all'attività, né all'uomo.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, è ormai unanimemente riconosciuto che la precocità della diagnosi, la qualità delle prestazioni erogate, la collegialità e la fattiva collaborazione dei vari operatori coinvolti - psicomotricisti, logopedisti, educatori socio-pedagogici - è fondamentale nell'ottenere i migliori e più evidenti risultati nel percorso riabilitativo dei bambini con spettro autistico. Ebbene, la Regione Campania ha deliberato un provvedimento che va esattamente nella direzione opposta: ha decretato un taglio alle ore (già poche, per la verità) di terapia cui ogni bambino autistico ha diritto. inoltre l'estromissione di alcune figure professionali, in particolare pedagogisti e operatori sociopedagogici, i quali fanno parte della squadra che prende in carico il bambino autistico e che partecipa attivamente al suo attivamente al suo progetto riabilitativo e al suo percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale. La vice presidente del Consiglio regionale della Campania, l'onorevole Valeria Ciarambino del MoVimento 5 Stelle, ha chiesto l'immediata sospensione di questa delibera, che offende, nella sua crudezza e nelle sue motivazioni prettamente collegate a risparmi economici, la dignità dei bambini autistici e delle loro famiglie. Voglio ribadire ancora una volta con forza che la battaglia per l'autismo si combatte con fatti e interventi concreti, non a parole o a passerelle. Parliamo di riduzione delle liste e dei tempi di attesa per l'accesso ai centri accreditati, che in qualche caso superano anche un anno. Parliamo del riconoscimento e dell'autorizzazione, da parte di ogni azienda sanitaria, ad adottare le migliori terapie scientificamente riconosciute, metodo ABA *in primis*, e del diritto di ogni piccolo paziente di poterne usufruire gratuitamente, indipendentemente dal luogo dove egli vive. Vi sono famiglie in condizioni economiche disagiate, le quali non possono accedere a queste terapie innovative. A tal proposito ho presentato un disegno di legge (Atto Senato 1397), che giace ancora in Commissione, e un emendamento al decreto-legge sostegni, purtroppo non approvato dal Ministero della salute, per cercare di ridurre queste vere e proprie gravissime sperequazioni. I bambini autistici vanno assistiti in maniera efficace e precocemente, per garantire loro un percorso riabilitativo capace di recuperare tutti i loro margini di autonomia. Essi hanno bisogno di un aiuto, non di rifiuti; non si può risparmiare sulla pelle dei bambini e degli adolescenti più fragili.

tutti noi abbiamo verso gli altri. Senza questo patto di fiducia non si può fare niente nella nostra società. Non si può prendere un aereo, se il patto di fiducia non sussiste, perché chiaramente, quando qualcuno di noi sale su un aereo, sta dando fiducia a chi quell'aereo l'ha progettato e l'ha costruito, a chi lo guida e a chi lo ha manutenuto e controllato. Allora, alla luce anche di tutte le cose che stanno succedendo negli ultimi tempi, vorrei fare un appello al Governo per questo decreto semplificazioni che sta arrivando. Se per velocizzare la nostra economia e semplificare si deve venir meno al controllo pubblico sulle azioni umane, noi mettiamo a rischio il patto

gravissimo, può essere enormemente grave. Abbiamo avuto 185 morti sul lavoro nel primo trimestre, ossia due morti al giorno dall'inizio dell'anno. Ho difficoltà a parlare della strage del Mottarone o del ponte Morandi, dove è stata la cattiva manutenzione a creare delle stragi. Noi dobbiamo capire in che direzione vogliamo andare, se vogliamo salvaguardare il patto sociale di fiducia o vogliamo che esso venga meno; con il sicuramente la ripresa socio-economica di questo Paese non ci sarà mai. Quindi, affinché le semplificazioni e le velocizzazioni non siano a discapito dei controlli e del controllo pubblico sulle operazioni private, io faccio un appello qui e ora al Governo, affinché il decreto in arrivo mantenga e ci assicuri i controlli necessari su tutte le operazioni che serviranno alla collettività. *(Applausi)*.

grazie a tutti

è stato modificato di comune accordo, grazie alla collaborazione del sottosegretario Scalfarotto, che ringrazio molto per la disponibilità e l'attenzione dimostrata, e di tutti i membri della Commissione. I punti fondamentali

si presenti alle elezioni comunali. Il *quorum* oggi è del 50 per cento per poter scongiurare il rischio di commissariamento

1 è il risultato dei lavori della Commissione ed è stato ripresentato come emendamento del relatore.

ogni candidato è comunque nella condizione di recuperare almeno una firma, che sia da un parente, da un amico o da un conoscente, per non andare proprio a penalizzare la raccolta firme nei piccoli Comuni.

L'articolo 60 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570,

prima in riferimento agli articoli 1 e 2, abbiamo presentato e votato in Commissione un emendamento di coordinamento per fare in modo che la legge, una volta arrivata nelle mani dei cittadini e ovviamente dei futuri candidati, sia la più chiara possibile, quindi abbiamo operato una rinumerazione

e la buona volontà che dimostrano nel candidarsi e continuare a lavorare in una situazione veramente difficile per tutti i nostri territori. Mi auguro dunque che quello di una serie di provvedimenti, anche puntuali come questo, visto che il loro *iter* procede più velocemente e trovano l'accordo di tutti, per migliorare le condizioni di lavoro nelle amministrazioni locali, perché è lì che c'è la politica con la P maiuscola

Signor Presidente, intervengo semplicemente per esprimere apprezzamento per il modo in cui si è lavorato in Commissione e nel comitato ristretto su questo testo. Il tema, come ha detto la relatrice, è - oserei dire - di democrazia reale in alcuni territori marginali, nei quali si verificavano purtroppo situazioni che non aiutavano le comunità locali

cioè che venivano da altre comunità a candidarsi in piccolissimi Comuni dove ce n'era una unica, in qualche misura per occupare gli spazi delle minoranze, creando una serie di problemi e di diseconomie locali: in questo caso, l'inserimento di un numero minimo di firme anche per i Comuni al di sotto dei 1.000 abitanti credo abbia bene affrontato e risolto la questione. La seconda questione è legata al raggiungimento del *quorum* laddove c'era un candidato unico, cosa che, nel combinato disposto della riduzione negli ultimi tempi del numero degli elettori in generale e di molti iscritti nelle liste dell'AIRE, di fatto era

tutte le persone che hanno contribuito e collaborato, *in primis* la relatrice, il sottosegretario Scalfarotto e tutti i membri della Commissione e del comitato ristretto, senza dimenticare gli uffici della 1a Commissione e del Ministero, che hanno dato un contributo importante; è bene ricordarsi anche di loro e del loro supporto,

sono anche o sono stati amministratori locali, quindi c'è una spiccata sensibilità per questo aspetto. Per il

Questa legge tratta, con due articoli diversi, due problematiche diverse, apparentemente sono disgiunte tra di loro, che in realtà si integrano e si sostengono a vicenda; c'è questo interscambio di utilità reciproca tra i due articoli e per questo è necessario che siano presenti nello stesso provvedimento. Il punto di partenza è stato quello di affrontare queste due tematiche specifiche, ma è anche stata la volontà di affrontare quello che sta diventando sempre di più un problema, ovvero la difficoltà di trovare persone disponibili permettetemi di usare questo termine - a sacrificarsi a volte per ricoprire il ruolo di sindaco nei piccoli Comuni. Le problematiche sono tante, a partire da un'indennità irrisoria

Il rischio di trovarsi con paesi, cittadine o piccoli Comuni commissariati è sempre più alto, perché, come tutti sappiamo, se l'elezione viene dichiarata nulla il Comune viene commissariato.

Vengono tolti dal *quorum* gli elettori residenti all'estero, iscritti al registro AIRE. Chiaramente non viene tolto loro il diritto di voto (ci mancherebbe, è sacrosanto); tuttavia, se

Faccio presente che in alcuni Comuni si arriva ad avere una percentuale di rappresentanza AIRE superiore al 50 ipotizzando un pieno sostegno all'unica lista di tutto l'elettorato dei residenti, l'elezione sarebbe comunque nulla. Spesso e volentieri, l'unica ancora di salvezza era proprio la seconda lista di di supporto, che permettesse di aggirare il raggiungimento del *quorum*. Da qui nasce il collegamento con il secondo articolo, che va a cercare di limitare

da svariate ragioni. La prima è quella, per certe categorie, di aver accesso a un periodo di aspettativa pari a quello della campagna elettorale: ci si regala un mese di ferie gratis, a spese del contribuente, senza avere alcun interesse per la tornata elettorale. La seconda categoria è costituita - come diceva il collega Taricco liste che arrivano da fuori, anche da fuori Regione, unicamente monitorando dove vi è una seconda lista, perché anche con pochissimi voti si riesce a essere eletti consiglieri comunali e quindi a godere dei permessi retribuiti per assenza dal lavoro e di *benefit* vari. Questo genera per quei piccoli - a volte micro - Comuni costi che diventano insostenibili. Il bilancio comunale, nella sua parte agibile, va tutto a coprire le spese che vengono generate da queste liste farlocche. Vi è poi una terza ragione, che è quella di una visibilità politica di alcune liste, magari anche aree estremiste (non faccio distinzione tra destra e sinistra), che, pur di avere qualche eletto, vanno a candidarsi e a presentarsi in paesini di montagna, per poi da lì agire politicamente. Chiaramente questo snatura e mette in seria difficoltà

Da ciò è derivata la scelta di inserire l'obbligo di presentare le firme dei sottoscrittori a sostegno delle liste anche nei Comuni sotto i 1.000 abitanti, che ne erano privi, unicamente perché serva a dimostrare che quella lista abbia un legame e una fiducia con Non aggiungo altro. Ovviamente, come si diceva prima, auspichiamo tutti che questa sera, in questo ramo del Parlamento, il disegno di legge venga approvato. Auspichiamo che ci sia una rapida seconda lettura, in modo da poter applicare la legge già nelle elezioni del prossimo autunno. Siamo consapevoli, per quanto ci riguarda, di aver svolto il nostro lavoro. Continueremo a farlo e a dare attenzione ai piccoli Comuni, soprattutto a quei 5.000 piccoli Comuni che sono l'ossatura del nostro Paese e che sono il *front desk* della pubblica amministrazione. nella stragrande maggioranza dei casi l'interlocutore diretto è il sindaco. Questo disegno di legge è anche un modo per dire grazie a tutti i sindaci per il lavoro che fanno e per la dedizione che ci mettono. Grazie, sindaci.

Ritengo che ogni dibattito e ogni intervento sui Comuni sia uno dei modi più efficaci per occuparci delle comunità che vi vivono. La valorizzazione delle nostre comunità territoriali per il tramite degli enti che li rappresentano, ne curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo era uno degli obiettivi della riforma del Titolo V che ha sovvertito la formulazione dell'articolo 114 della Costituzione. Pensate che siamo passati dall'originaria formulazione, che ripartiva la nostra Repubblica in Regioni, Province e Comuni, attuale, che ha stabilito che la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. Come vedete, il cambio di paradigma è netto. La nuova formulazione attribuisce massimo valore agli enti di maggiore prossimità ai cittadini e dà concreta attuazione al precetto di cui all'articolo 5 della Costituzione. Inoltre, questa norma costituisce la base per il principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 118 della Costituzione, che assegna le funzioni amministrative in via principale proprio ai Comuni. Il descritto impianto definito dalla nostra Carta costituzionale dovrebbe già far comprendere l'importanza dei temi trattati oggi. Il discorso è valido ancora di più considerando che il disegno di legge in discussione riguarda anche la materia elettorale. Solo qualche settimana fa, in occasione dell'*iter* di conversione in legge del decreto che ha differito le elezioni amministrative previste per questa primavera all'autunno prossimo, è stato approvato un emendamento da me presentato che, per la prima volta, permette di inviare le nomine dei rappresentanti di lista tramite posta elettronica certificata ed evitare l'autenticazione della firma del delegato qualora l'atto sia stato firmato elettronicamente dal delegato stesso. la misura è stata prevista per la tornata elettorale del prossimo autunno, ma l'Assemblea ha già dato prova di mostrarsi sensibile all'obiettivo di semplificare e digitalizzare i procedimenti elettorali. A tal proposito, desidero ringraziare tutti i senatori che hanno sottoscritto il mio disegno di legge, attualmente all'esame della Commissione affari costituzionali, che mira a dare stabilità alla misura a tutti i livelli territoriali ed elettorali. Non meno importante è il disegno di legge che oggi ci apprestiamo ad approvare. L'intervento normativo interviene sulla legge n. 81 del 1993, prevedendo un numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati al Consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco nei Comuni più piccoli. Al contempo, si interviene sul testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali riducendo al 40 per cento il *quorum* strutturale richiesto per la validità delle elezioni amministrative nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Nel computo, peraltro, non si terrà conto degli elettori iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero che non hanno votato. Si tratta di modifiche tecnicamente semplici, ma destinate a semplificare la normativa elettorale dei piccoli Comuni ed evitare che gli stessi vengano paralizzati a causa del numero di residenti che si trovano impossibilitati a esercitare il diritto di voto perché fuori sede o residenti all'estero. Si tratta di un altro piccolo tassello che va a comporre un mosaico ben più ampio, quello di tutte le riforme epocali che, anche grazie al MoVimento 5 Stelle, sul pezzo da anni, siamo riusciti ad approvare nelle corso di questa legislatura, mentre altre sono *in itinere*. Il nostro Paese attendeva tali riforme da decenni e neanche la brusca interruzione dei due Governi presieduti dal nostro Giuseppe Conte è riuscita ad arrestarle. In quel caso, a vincere furono il trasformismo e i giochi di palazzo, che sicuramente non interessano tutti i cittadini che si trovano oggi fuori da quest'Aula; oggi, invece, sono proprio loro a vincere, soprattutto coloro che vivono nei piccoli Comuni, realtà modeste e spesso periferiche che meritano di essere valorizzate e sostenute da tutti noi.

parere sull'emendamento 1.100 è contrario.

che l'articolo 1 prevede l'abbassamento del *quorum* nel caso in cui venga presentata una sola lista. Questo non è un tema che vuole semplificare le elezioni di un sindaco; meglio, vuole far quello perché in molti casi, laddove non si trovano delle candidature e non si riesce a creare una contrapposizione tra due o più liste, vi è la necessità di salvaguardare la possibilità che anche una sola lista possa portare all'elezione del sindaco, riducendo il *quorum* di partecipazione. Prima era del 50 per cento, ora viene spostato al 40, sottraendo agli iscritti i residenti all'estero iscritti all'AIRE che non partecipano al voto, così consentendo di sottrarre quei Comuni dal possibile commissariamento. Avere un commissario o avere un sindaco, infatti, non è la stessa cosa, come sanno bene i cittadini che si trovano nelle condizioni di doversi rapportare con un commissario e non con un sindaco. Il secondo articolo, relativo alle firme di sottoscrizione delle liste, va ugualmente nella direzione di consentire l'abbassamento del numero delle firme necessarie,

nei Comuni con un numero di abitanti inferiore a mille, non era necessario presentare firme di sottoscrizione. Di fatto si rafforza un principio democratico, perché evita la possibilità che arrivino all'ultimo minuto, come avviene normalmente, liste costruite in altri territori solo per marcare una presenza. In tal modo, mettendo un numero simbolico di 5-10 firme, si evita di sottrarre totalmente a quella comunità la possibilità di esercitare democraticamente un controllo anche sulla presentazione delle liste, prevedendo quindi un minimo di firme possibili. È un provvedimento su cui non bisogna dire molto altro. Va valorizzato lo spirito che ci ha portato ad essere insieme nella definizione di queste norme, perché, quando si parla di enti locali, deve esserci la necessaria deve esserci la necessaria volontà di trovare soluzioni comuni. Oggi vediamo come il mestiere del sindaco sia quello più complesso.

Grazie a tutto

riteniamo si tratti certamente di un provvedimento migliorativo, di un passo in avanti rispetto ad un problema che abbiamo segnalato anche noi da diverso tempo. Non lo reputiamo ottimo, perché a nostro giudizio sarebbe stato molto più semplice e lineare, come proponeva in origine anche l'ANCI, prevedere la soglia dei voti riportati al 20

un compromesso accettabile quello che è stato trovato e ci permettiamo, in questa sede, dove l'analisi tecnica all'articolo di richiamare l'attenzione del Governo e di tutte le forze politiche ai problemi che vivono i cittadini delle comunità più piccole, soprattutto quelle delle aree interne, che soffrono di un problema di

di perdere tanti Comuni, tante identità, tante ricchezze che rappresentano l'anima della nostra Nazione. Rivolgo

alcuni aspetti riguardanti le prossime elezioni che, a nostro avviso, non avrebbero dovuto essere rimandate. Non si può, infatti, mandare in *lockdown* anche la democrazia, visto che si è votato in tutte le realtà europee; realtà alle quali molto spesso vi richiamate. Solo in Italia questo non è stato possibile e aspettiamo ancora una data individuata all'interno della finestra. Speriamo che la decisione possa essere presa al più ma certamente senza alleggerire nella maniera più assoluta - e lo diciamo da destra, da partito della legge della legge - le procedure che certificano la moralità dei candidati. Procedure che avrebbero dovuto essere alleggerite anche alla luce delle condizioni in cui versano ancora gli uffici pubblici. Voglio ringraziare la Commissione, la relatrice, il gruppo di lavoro per questo che riteniamo un passo avanti, e confermo il voto favorevole di Fratelli d'Italia.

che solitamente usiamo definire piccoli Comuni. Questi Comuni non rappresentano soltanto una fetta consistente e numericamente importante nel novero complessivo di tutti i Comuni italiani, ma rappresentano qualcosa di più, sia nella storia sociale e civile del Paese sia - credo - nel futuro diverso che oggi, dopo oltre un anno di pandemia, possiamo e dobbiamo immaginare. Su questo obiettivo il Partito Democratico c'è sempre stato e sempre continuerà a esserci. Ecco perché abbiamo lavorato a questo provvedimento nell'obiettivo di rendere

particolarmente l'incidenza degli iscritti all'AIRE per raggiungere il famoso *quorum* nel caso di una sola lista. La seconda questione concerne le liste opportunistiche e strumentali che vengono da fuori del territorio del singolo Comune. Il merito di entrambi i problemi è stato già chiarito. Voglio aggiungere solo due considerazioni: la prima riguarda le crescenti oggettive difficoltà che molti Comuni da tempo esprimevano, da ben prima che scoppiasse l'emergenza pandemica. Queste difficoltà sono legate soprattutto allo spopolamento diffuso che investe da tempo tempo le aree più periferiche del nostro Paese. È un fenomeno profondo che ha radici sociali ed economiche che non possono essere risolte intervenendo solo ed esclusivamente sulle regole. È chiaro, poi, che, tra i molti effetti che lo svuotamento di questi centri produce, c'è anche una partecipazione, purtroppo, sempre più limitata alla vita pubblica, quindi anche al voto da parte degli aventi diritti, siano essi residenti sia, in misura maggiore, gli iscritti all'AIRE. Sul tema degli iscritti all'AIRE, soprattutto nei Comuni più piccoli, parliamo molto spesso di persone che non esercitano più il diritto di voto da tempo, con la conseguenza possibile ma effettivamente concreta - di contribuire a rendere invalida l'elezione per mancato raggiungimento del *quorum*. A tutto questo possiamo e dobbiamo dare una soluzione che tuteli sostanzialmente tre elementi: validità delle elezioni, principio democratico e piena legittimazione elettorale degli organi rappresentativi. La seconda considerazione riguarda l'aspetto più strettamente costituzionale di questo disegno di legge, che è legato soprattutto a due profili: da un lato, la soglia più bassa definita per il *quorum*, che passa da 50 a 40 per cento; dall'altra, il tema degli iscritti all'estero, quindi il rapporto tra cittadinanza e residenza per il voto nelle elezioni locali, che è la cornice in cui si inserisce ogni valutazione sullo scorporo dei cittadini iscritti all'AIRE. Se il diritto di voto dall'estero non è previsto per le elezioni locali, come invece lo è per le elezioni politiche generali e per i *referendum*, le ragioni sono chiare. C'è senza dubbio una motivazione legata all'importanza specifica del radicamento territoriale in questo tipo di elezioni e l'esigenza che l'elettore dimostri questo radicamento con la presenza diretta alle elezioni. Ripeto che tutto questo è chiaro e ben comprensibile, ma si accompagna con l'esigenza di evitare distorsioni per quanto riguarda la validità di un'elezione, nel caso in cui si presenti una sola lista. In questa direzione, per evitare possibili distorsioni, va scelto di scorporare dal computo del *quorum* gli elettori residenti all'estero. Questo per dire che quella odierna non è una soluzione nuova per il Partito Democratico, che invece è stato tra i primi, in passato, a presentare proposte di legge simili. Si tratta dunque di una proposta che oggi non possiamo che giudicare equilibrata dal punto di vista dei principi costituzionali e capace di dare risposte che, da tempo, Comuni italiani (ANCI) e i loro rappresentanti, chiedono. Aggiungo infine una parola sull'estensione delle sottoscrizioni delle liste per i Comuni tra i 2.000 e i 500 abitanti, per evitare che si approfitti della riserva elettiva a garanzia delle minoranze, da parte di liste che nascono con obiettivi che sono abbastanza lontani dal bene di una comunità e di un territorio. È stato osservato, anche in modo comprensibile, il rischio che l'introduzione delle delle firme possa rivelarsi un ostacolo, anziché una tutela per la presentazione dei candidati. Capisco l'osservazione, ma credo che anche il pericolo di effetti controproducenti possa essere escluso, così come previsto dalla diversa modulazione del numero di firme proporzionali agli abitanti. mi auguro davvero che il provvedimento in esame sia il primo concreto passo per rispondere ai nodi che restano aperti per tanti piccoli Comuni: penso ad esempio al riconoscimento di un'indennità congrua ai sindaci, al tema della gestione associata, così come alla questione del superamento dei limiti di mandato. Anche dalle risposte a questi temi passa il rafforzamento necessario di una parte imprescindibile della struttura sociale e amministrativa del nostro Paese. Per tutte queste ragioni, quindi per il merito del provvedimento finale e perché abbiamo contribuito a questo testo condiviso, il voto del Partito Democratico sul disegno di legge in esame Dichiaro chiusa la votazione per l'elezione di due senatori Segretari. Invito i senatori Segretari a procedere allo spoglio delle schede.

Il lavoro fatto ci permette di arrivare all'approvazione del disegno di legge, grazie anche alla disponibilità, alla collaborazione e al lavoro

molto spesso condizioni non semplici e di disagio, ad esempio dal punto di vista dei servizi, dei trasporti e delle comunicazioni. Vorrei ricordare che nella scorsa legislatura è stata approvata una legge molto importante,

non si tiene conto degli elettori iscritti all'AIRE: questo è fondamentale proprio per i ragionamenti che facevo prima. Sappiamo infatti quello che avveniva: molto spesso si facevano delle liste quasi

considerata inutile, perché si dà per scontato la vittoria. Intervenire sul *quorum* è quindi fondamentale, eliminando gli iscritti non votanti: questo è assolutamente importante.

e ridare forza al momento delle elezioni democratiche. Essere intervenuti con l'articolo 2 per fare in modo che

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, non voglio soffermarmi sul merito di questo provvedimento. Ho partecipato al comitato ristretto, i colleghi l'hanno illustrato, la relatrice è stata puntuale e i colleghi che mi hanno preceduto hanno ripetuto tutti i passaggi che ci hanno portato a licenziare questo testo. A me piace, in questa sede, parlare del metodo,

con i rappresentanti di tutti i Gruppi, che approfondiscono una singola materia, si arriva a posizioni condivise. Alla fine, infatti, chi fa politica, chi fa le liste, chi presenta le candidature sa quali sono i problemi

che metta da parte le contrapposizioni e le diversità e si faccia corpo unico nei confronti degli interessi reali del Paese, in questo caso dei piccoli Comuni e degli amministratori, che chiedevano da tempo che si intervenisse su questa materia.

tematiche. È la politica dei piccoli passi, di quelli che servono. Oggi abbiamo incardinato il disegno di legge Lanzi, che vuole stabilizzare una norma che era stata già approvata

le elezioni amministrative, di acquisire i certificati penali. Questo è il modo di fare politica: lasciamo da parte i grandi temi che ci possono separare. Questa è una maggioranza

un modo corretto di operare, che ci fa ritenere la nostra missione realizzata in pieno. Quando torniamo nei nostri territori, guardandoci allo specchio, possiamo dire: abbiamo dato un contributo a migliorare una certa situazione. In questa circostanza l'abbiamo fatto; la Commissione affari costituzionali lo ha fatto in precedenza, con altri provvedimenti, e si appresta a farlo per altri ancora. Se questa è la filosofia che tutto il Parlamento assumerà come punto di riferimento, credo che alla fine di questa legislatura - qualunque sarà il momento

Con le misure contenute nei due articoli, già illustrati dalla relatrice Pirovano, eviteremo il commissariamento soprattutto nei piccoli Comuni.

consenso fanno la guerra al candidato sindaco e alla lista unica scoraggiando le persone ad andare a votare. Ciò è uno sbaglio enorme. Chiunque sia il candidato, di qualunque corrente politica (da destra a sinistra), se c'è una sola lista è giusto che quel candidato e quell'amministrazione vengano votati. Chi scoraggia la gente ad andare a votare

sindaci che quotidianamente portano gli anziani, con l'auto dei servizi sociali, nei CEOD, nei centri di sostegno e negli ospedali e che fanno attraversare i bambini sulle strade davanti alle scuole. Sono sindaci tuttofare che spalano la neve, tagliano l'erba e fanno tante altre cose di ordinaria amministrazione che, a livelli superiori della politica, anche per una questione di tempo, non si fanno. Sono persone che amano la propria comunità. La Lega è vicina ai sindaci. Viva i sindaci d'Italia e soprattutto quelli dei piccoli Comuni. Ringrazio la Commissione per i lavori svolti sul provvedimento

in particolare delle Forze di polizia, che, visto che la legge lo permette, presentano una lista alternativa a quella del sindaco pur di avere un'aspettativa temporanea per la campagna elettorale. Riporto l'articolo: passione per la pubblica amministrazione, per la politica, voglia di staccare dal lavoro quotidiano per un periodo (peraltro retribuito), o è solo una coincidenza quella che vede una quarantina di dipendenti pubblici candidati alle elezioni comunali del prossimo 10 giugno? tutti Comuni piccoli, in cui non è necessario raccogliere firme per presentare una lista. Nel nostro caso stiamo parlando di San Mauro di Saline e Borgofranco sul Po, in provincia di Mantova.

del nostro Paese. Lo stesso è accaduto per un'altra lista a San Mauro di Saline, in provincia di Verona. Quello delle aspettative elettorali è un fenomeno nato in sordina una decina di anni fa, ma che è andato via via crescendo fino ad assumere proporzioni considerevoli.

(il Veneto ha dato un forte contributo all'emigrazione in quel periodo).

all'estero. Nel mio Gruppo politico, che conosco molto bene, abbiamo fatto la gavetta masticando pane, territorio e amministrazioni locali. Questa è la nostra storia. Nel nostro *curriculum* vantiamo un cammino che parte proprio dai Comuni, le fondamenta della politica italiana. Per questo, quando i miei colleghi della Commissione affari costituzionali si rivolgono a voi, colleghi,

non ha una storia basata sui Comuni, sui sindaci e, non conoscendo le problematiche delle piccole comunità,

che reca importanti migliorie in termini di elezioni comunali. Nel corso degli anni sono emersi in questo ambito problemi che il legislatore ha deciso di risolvere attraverso il provvedimento Il primo problema riguardava la validità stessa delle elezioni. La norma vigente prevedeva che qualora alle elezioni comunali fosse stata ammessa un'unica lista, la consultazione sarebbe stata valida solo nel caso in cui il numero dei votanti non fosse inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune. La norma in questione ha generato diverse complicazioni, in particolar modo nei Comuni più piccoli, massicciamente interessati da fenomeni di emigrazione di massa. È noto, infatti, che coloro che si sono trasferiti all'estero restano iscritti nelle liste elettorali del Comune di ultima residenza. Tali elettori lontani dall'Italia, che spesso non conoscono le situazioni del loro Paese d'origine, pur non essendo, come detto, iscritti alle liste elettorali, generalmente non esercitano il voto e possono far mancare il *quorum* di validità della consultazione. La questione concernente il computo degli elettori emigrati all'estero, nel caso di votazioni per le quali è previsto un *quorum* strutturale, non è per la verità affatto nuovo: in occasione del voto referendario del 2000 sul Titolo V, si pose con asprezza di toni il problema di alcune centinaia di migliaia di cittadini trasferitisi all'estero che, pur risultando iscritti, erano da anni irreperibili e contribuivano quindi di fatto a innalzare il *quorum* di validità del *referendum*. Ancora in occasione del *referendum* sulla procreazione medicalmente assistita del 2005, i promotori hanno fatto inutilmente notare le pesanti discrepanze tra il numero degli italiani residenti all'estero cui è riconosciuto il diritto di voto ai fini del calcolo del *quorum* strutturale e il numero di coloro che risultavano effettivamente reperibili. A tal fine, la norma approvata in Commissione prevede di escludere gli elettori iscritti all'AIRE che non hanno votato. L'elezione, ove sia stata ammessa una sola lista, è valida purché abbia riportato un numero di voti validi inferiore al 50 per cento e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti alle liste elettorali. È bene ricordare che rimane garantita al cittadino residente all'estero che si presenti il giorno delle elezioni comunali nella sezione elettorale a lui assegnata, la facoltà di esercitare liberamente il proprio diritto elettorale. Quindi non c'è nessuna violazione dell'eguaglianza del voto o una qualsiasi preclusione per i nostri concittadini all'estero. Il secondo intervento va ad incidere, invece, sul numero di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste di candidati al Consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco. Il testo approvato in Commissione è frutto di un confronto tra le forze politiche che ha consentito di ottenere una sintesi efficace tra l'esigenza di rapportare il numero delle sottoscrizioni a quello degli abitanti per non penalizzare i Comuni più piccoli e quella, nel contempo, di scoraggiare la presentazione di liste totalmente disgiunte dal territorio. Ritengo, colleghe e colleghi, che con questo provvedimento si possa favorire un ordinamento degli enti locali che tenga conto della modernità e delle esigenze del territorio, un sistema che guarda al futuro. E per futuro intendo più sinergie tra i Comuni più piccoli per affrontare difficoltà simili, quindi maggiori fusioni per migliorare i servizi alla cittadinanza. Questo provvedimento può essere un passo anche in tal senso. In conclusione, annuncio il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle.